05/06/2024); Presidente del Consiglio dei ministri Ministro della salute Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi

dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa* della difesa* «Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile

in seduta comune è convocato martedì 25 giugno alle ore 12,30 per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

una dipendente del Senato venuta a mancare dopo una lunga malattia lo scorso 5 giugno, all'età di 58 anni. Si tratta della dottoressa Maria Maddalena Fischetti.

per la sua disponibilità e il suo tratto umano garbato e cordiale. Siamo vicini alla famiglia, al marito Carmelo, ai figli Martina e Simone, ai quali va la sentita partecipazione di tutto il Senato che per qualche secondo la ricorda in

Benché non sia iscritto all'ordine del giorno, ho piacere di dare

tutti conoscete: parlo di Enrico Berlinguer. Abbiamo stabilito che parli solo il rappresentante del Gruppo al quale apparteneva, così come faremo domani,

il cuore di Enrico Berlinguer cessava di battere. La sua morte, per tanti motivi, ha segnato uno spartiacque nella storia della nostra Repubblica. Berlinguer era amato e rispettato, al di là delle appartenenze politiche, per la sua etica, per il suo carisma profondo, per la dolcezza del suo sguardo. Il suo nome, Berlinguer, così difficile da pronunciare, divenne un amuleto per milioni di persone, soprattutto le più semplici e le più indifese. La sera del 7 giugno un malore lo aveva colpito sul palco di Padova, durante un comizio elettorale, in mezzo ad una piazza piena di popolo. Per quattro giorni l'Italia intera stette come sospesa, in attesa di un miracolo: che Berlinguer potesse riaprire i suoi occhi e il suo sorriso che appartenevano ad un popolo intero che in lui si identificava, così come Berlinguer aveva scelto di appartenere ad un popolo, di stare da una parte della storia, quella degli ultimi, di chi è più debole, di chi reclama diritti ed emancipazione. Berlinguer, di famiglia borghese, decise giovanissimo di diventare comunista perché convinto dalle argomentazioni di operai, manovali e artigiani antifascisti che frequentava di nascosto in una stalla nelle campagne intorno alla sua Sassari. Nel gennaio del 1944, nei giorni più duri dell'inverno e della fame, organizzò con altri giovani una manifestazione per chiedere farina e pane per la sua popolazione. Venne incarcerato per cento giorni. Berlinguer fu questo: per tutta la sua vita fu tutt'uno con le istanze di un popolo da riscattare, che fece coincidere con le istanze della Repubblica e della democrazia appena nate, da conquistare, da rafforzare e da difendere ogni giorno innanzitutto nell'incontro e nell'unità delle masse popolari. Berlinguer, da comunista, volle sempre, testardamente, l'incontro con i cattolici, con la cultura e i valori del cristianesimo. Le sue mani e quelle di Aldo Moro che si stringono insieme sono una delle immagini più belle della nostra Repubblica. Quando il terrorismo e gli apparati deviati uccisero Moro, morì una prima volta anche Berlinguer. E venne fermato per sempre il più grande tentativo di cambiamento. Berlinguer fu il *leader* comunista che affermò il valore assoluto, imprescindibile e universale della democrazia e la possibilità di costruire socialismo solo nella democrazia e nella libertà. unì nella sua persona il portato della generazione dei partigiani che avevano consegnato all'Italia la libertà e lo slancio di futuro delle generazioni che generosamente stavano costruendo la Repubblica. Per questo in Italia la parola "comunista" ha un valore alto e unico. Fu europeista convinto; e in quella campagna per il Parlamento europeo del 1984 chiese ad Altiero Spinelli di candidarsi come indipendente con il Partito comunista. La parola "pace" fu quella più pronunciata da Berlinguer in quella sua ultima campagna elettorale. Sul palco di Padova volle a tutti i costi finire il suo discorso e le sue ultime parole furono per "l'Italia" dei giovani e "delle donne che vogliono cambiare la società". E quando il feretro di Berlinguer arrivò a Roma, un corteo infinito lo accompagnò per l'ultima volta in Piazza San Giovanni. un popolo intero, con le sue ferite e con le sue battaglie; metalmeccanici, braccianti, le donne indomite delle baracche delle periferie urbane, le donne irpine e lucane con le quali aveva sostato a lungo dopo la notte del terremoto del 23 novembre 1980. Fu dopo quella notte che Berlinguer decise che era urgente un tempo di nuove battaglie sociali. In quel corteo infinito, Presidente, di bandiere rosse, di pugni chiusi, di lacrime, di gonfaloni dei Comuni, di persone arrampicate di persone arrampicate sugli alberi e sui cornicioni per chiamare ancora una volta il suo nome, c'era, tra tutti, Sandro Pertini, il Presidente partigiano, che si inginocchiò davanti al feretro, lo baciò e si strinse alla folla. C'era un popolo intorno a Berlinguer. La diversità di Berlinguer non fu mai isolamento; è la diversità di chi non si vuole arrendere ad un mondo ingiusto, fatto per pochi, fatto di diseguaglianze e di privilegi. La questione morale in Berlinguer è tutt'uno con la questione sociale, di riscatto e di speranza; ed è quanto mai urgente, adesso, nel tempo che viviamo. *(Vivi,

Benché avessimo previsto un solo intervento, credo che il Gruppo Misto, che me lo chiede con insistenza, abbia eguale diritto di discendenza. Quindi diamo al senatore Magni la parola per cinque minuti.

militavo in quel partito. Vorrei sottolineare che nel 1973, a fronte del golpe del generale Pinochet Berlinguer annunciò una svolta del Partito Comunista Italiano. Affrontò la questione del compromesso storico, cioè il ragionamento in cui diceva che, in sostanza, da quel momento era necessario che la cultura cattolica, la cultura socialista e quella comunista trovassero un grande

nel nostro Paese; egli con grande coraggio affrontò questo tema, che non fu per niente facile, neanche all'interno del suo stesso partito. Questo è stato un momento importante. Un altro momento importante è

e aprendo un confronto diverso. Vorrei sottolineare anche la specificità di un comunista italiano che sostanzialmente era un grande democratico del nostro Paese. Infine, per farla breve, la battaglia del 1984 sui quattro punti di taglio della scala mobile. Noi affrontammo e avemmo di fronte un partito che si divise, anche a sinistra; lo stesso sindacato e via dicendo. facemmo una battaglia in cui il sostegno di Berlinguer ai lavoratori fu determinante, ma perdemmo il referendum. Vorrei ricordare che il referendum lo sostenevamo noi del Partito Comunista, Comunista, la CGIL e l'MSI; vorrei sottolineare il dato anomalo di quella battaglia. Sono stati tre momenti importanti, che ho vissuto personalmente da militante e da partecipante iscritto a quel partito, dentro il movimento sindacale.

È stato un momento importante, questo del ricordo di Enrico Berlinguer, che voglio ricordare anch'io. A Padova, quarant'anni fa, concluse il suo intervento elettorale, benché già colpito visibilmente dall'ictus, quasi come un suo ultimo omaggio alla politica, alla quale credeva come soluzione dei problemi, di tutti i problemi. Io ricordo benissimo ahimè, ho l'età per ricordarne le tappe - che non è stato necessario che passassero gli anni (guardate che questa è una caratteristica che accomuna pochi) perché vi fosse una sorta di larga commozione pluripartisan. La commozione pluripartisan per Enrico Berlinguer ci fu subito, immediatamente. Non ho bisogno di testimoniare che anche il mio capo politico di allora vi partecipò, ma vi parteciparono italiani di tutte le fedi politiche, perché convinti, al di là delle sue idee, della linearità della sua coerenza, della sua onestà e del suo spendersi, anche a volte in conflitto con la sua tradizione politica,

C'è stata poco tempo fa una mostra di Sposetti, ci sono molti docufilm, il Partito Democratico gli ha dedicato la tessera, se non vado errato, per decisione della segretaria Schlein e c'è stata persino - ero presente anche in quella occasione - una *standing ovation* nella sede meno prevedibile, quella dei più lontani politicamente dalla sua storia politica. Questo aiuta ad immaginare sempre, nel ricordo di Enrico Berlinguer, che si possono contrastare le idee, ma bisogna sempre riconoscere la natura degli uomini che valgono e il cui ricordo rimane. Vi invito ad osservare

La Conferenza dei Capigruppo, che si è riunita il 29 maggio, ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 18 giugno. Questa settimana, con sedute senza orario di chiusura, proseguirà

la discussione del disegno di legge per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati. L'ordine del giorno di martedì 18 giugno, alle ore 16, prevede l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi questa settimana. Alcuni Capigruppo mi hanno già fatto pervenire una richiesta di convocazione della Conferenza dei Capigruppo, che fisso sin d'ora per domani alle ore 13.

per cui noi chiediamo di votare il calendario con delle proposte di modifica. Le proposte di modifica riguardano l'orario di fine chiusura delle sedute di questa settimana, che vorremmo fissare alle ore 20, nelle giornate di oggi, domani e giovedì.

grazie.

Signor Presidente, riprendendo la proposta del presidente Patuanelli, faccio notare a tutte le colleghe soprattutto dei Gruppi di maggioranza che, siccome entriamo nella fase centrale del provvedimento di riforma costituzionale, in particolar modo ripartendo dall'articolo 5 5 che riguarda l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, è evidente che questo articolo necessita non solo del tempo adeguato, ma anche della possibilità per i diversi Gruppi di avere maggior tempo a disposizione, che intanto si è esaurito per effetto dell'attivazione della tagliola. tagliola. Signor Presidente, come abbiamo già detto la settimana scorsa, questa settimana era caratterizzata da un provvedimento legato all'intelligenza artificiale, la che è stato discusso in 1a Commissione. Sarebbe quindi opportuno - vedo il presidente Balboni - evitare inutili sedute notturne della Commissione affari costituzionali, che si ritroverebbe a farle a farle se ci fosse una forzatura sui tempi dell'Assemblea. Penso di interpretare anche il volere degli altri Gruppi di opposizione dicendo che abbiamo già dato la nostra disponibilità nell'ultima Conferenza dei Presidenti

prima del G7 di porre sul tavolo dei Grandi anche questo provvedimento, indipendentemente dalla valutazione di merito che noi diamo (che probabilmente non è positiva). Indipendentemente dalla valutazione che esprimeremo in Commissione e in Aula, riteniamo doveroso da parte delle opposizioni non frenare il provvedimento.

Immagino che lei lo starà facendo pensando che questa nostra disponibilità sia condizionata dal lavoro che abbiamo sottolineato. In realtà lo dico davvero con senso di responsabilità. Lo avremmo fatto comunque affinché, di di fronte ai grandi della Terra, la Presidente del Consiglio possa porre le sue proposte sul tavolo, indipendentemente dalle valutazioni di merito anche delle opposizioni, che ovviamente non faranno sconti, ma saranno assolutamente costruttive. Detto questo, signor Presidente, le chiederemo anche un aggiornamento su alcune valutazioni che lei aveva rinviato

Signor Presidente, uniformandomi alle osservazioni formulate dai Capigruppo che hanno appena parlato, circa l'esigenza di procrastinare l'esame del provvedimento sul premierato, che non ha una scadenza contingente e che non è legato ad alcun aspetto di natura congiunturale immediata, vorrei richiamare alla sua attenzione ed all'attenzione dell'Aula una lettera che le ho inviato in data 4 giugno, che è il motivo della proposta che avanzo oggi, che è legata ad alcune circostanze che si stanno sviluppando nel corso di questa e delle prossime settimane, che attengono a momenti particolarmente importanti e significativi della nostra vita internazionale, della presenza del nostro Paese all'interno dei consessi internazionali, e che si stanno sviluppando senza che il Parlamento ne abbia discusso e abbia affidato un mandato al Governo in questa direzione. Mi riferisco, in particolare, alla cosiddetta Conferenza di alto livello per la pace in Ucraina, che si terrà nei prossimi giorni, il 15 e il 16 giugno, in Svizzera. in Svizzera. Come ha ricordato il presidente Boccia, ricordo che anche in una mia precedente asserzione in questa sede avevo chiesto uno specifico dibattito attorno ai temi dell'intelligenza artificiale, in connessione con lo svolgimento del

della questione ucraina, ma il Parlamento non ha dato alcun mandato al Presidente del Consiglio per muoversi in questa direzione. Infine, ma non meno importante, è stata fissata è stata fissata l'Assemblea del vertice della NATO a Washington per i prossimi 9 ed 11 luglio. È un tema su cui ci siamo lungamente profusi in sede pubblica. L'Assemblea parlamentare della NATO nei giorni scorsi a Sofia ha deliberato. Cosa farà il Governo in quella circostanza? Noi pensiamo che il Parlamento debba discutere una mozione e dare degli indirizzi al Governo in questo senso e crediamo che tutti questi aspetti siano più cogenti e siano più urgenti rispetto alla prosecuzione, in questa sede oggi, sede oggi, della discussione sul premierato. Quindi, sento di dover appoggiare l'istanza che è stata avanzata dai colleghi e chiedo che il calendario venga riformulato e rimodulato nei termini che hanno avanzato nelle loro richieste i presidenti Patuanelli e Boccia, oltre che con la nostra richiesta che ho appena espresso.

Presidente, intervengo per appoggiare, naturalmente, la proposta del nostro presidente Patuanelli, poi perfezionata anche dal presidente Boccia,

Aula. Ciò andrebbe anche incontro alla Conferenza dei Capigruppo da lei poc'anzi annunciata per le ore 13 di domani, che è destinata proprio a rivedere, ristabilire e rimodulare eventualmente i termini e i modi in cui la discussione sulla riforma costituzionale del premierato possa andare avanti. Mi sembra molto coerente, in questo progetto, fermarsi un attimo per consentire alle Commissioni di lavorare e quindi procedere in questo modo. Oltretutto, signor Presidente, faccio presente a lei, ma a tutta l'Assemblea, che è vero che non è materia di dibattito di questa Assemblea ma della Conferenza dei Capigruppo, che davvero il contingentamento voluto dalla maggioranza rispetto ai tempi di discussione della modifica costituzionale del premierato è è insopportabile e rimarrebbe come una macchia su questa maggioranza. Mi pare che il confronto democratico sia un valore che dovrebbe essere apprezzato da tutti e quindi mettere la mordacchia alle opposizioni per arrivare al traguardo - non si sa bene per quale motivo - entro il 18 giugno, quando non c'è una scadenza, quindi senza consentire un reale confronto all'interno dell'Aula,

piccolo *lapsus* prima, quando ha parlato di Enrico Berlinguer come componente del Gruppo del Partito Democratico. Questa è una bestemmia storica per ovvie ragioni, ma soprattutto perché

che non sia ossequiosa al Regolamento. Comunque, per sua conoscenza, la informo che al momento abbiamo già dedicato trentasette ore di dibattito a questa riforma, che sicuramente ne avrà almeno altre dieci o quindici,

molto più ampia, che toccava molti più articoli, ma non meno importante (o forse meno importante, a seconda delle valutazioni). Questo non ha importanza, comunque, riguardo

parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

Signor Presidente, iniziamo a trattare uno degli articoli più significativi della proposta di riforma. Iniziamo infatti a discutere dell'articolo che prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e la contestuale elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Non solo la riforma prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e la contestuale elezione delle Camere, ma prevede anche che sia assegnato su base nazionale un premio alle liste collegate al Presidente del Consiglio, che sia tale da garantire una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere. definisce i tratti salienti della riforma perché prevede l'elezione diretta, la contestuale elezione delle due Camere e l'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste collegate,

per la prima volta nel nostro ordinamento - e direi per la prima volta, guardando agli altri ordinamenti costituzionali vigenti o a quelli che la storia ci presenta - un inedito. Per la prima volta infatti noi eleggeremo due Assemblee parlamentari per trascinamento, in conseguenza dell'elezione del Presidente del Consiglio. Le Camere non saranno cioè più composte in base ai risultati elettorali relativi alle stesse Assemblee, non sarà più il voto diretto dei cittadini alle liste e ai candidati alle due Assemblee a determinare la composizione delle stesse.

In questo meccanismo che, ripeto, non ha eguali in nessun ordinamento costituzionale vigente si consuma la sottoposizione, la subordinazione del Parlamento al Presidente del Consiglio. E si consuma altresì quel ribaltamento del rapporto tra Parlamento e Governo che caratterizza invece la nostra forma di governo parlamentare e tutte le forme di governo parlamentari esistenti in Europa. Io non so se i colleghi che non hanno partecipato ai lavori della Commissione sono consapevoli di ciò che si apprestano a votare. Temo che non lo siano e devo dire che sono anche colpito dalla disattenzione e dal disinteresse con il quale noi in quest'Aula stiamo discutendo di una riforma così importante e così gravida di conseguenze per la nostra democrazia. Infatti, nello stravolgimento del rapporto tra Parlamento e Governo e in questa modifica della natura del Parlamento, si consuma una trasformazione della natura della democrazia pluralista, così come è stata faticosamente conquistata all'indomani del secondo conflitto mondiale. Stiamo cioè discutendo di un aspetto assolutamente fondamentale del nostro ordinamento costituzionale. Non si tratta di una riforma che opera una qualche manutenzione o che incide su aspetti marginali, ma di una riforma che stravolge in maniera radicale le caratteristiche della nostra democrazia perché il Parlamento non sarà più espressione del pluralismo politico e sociale, non sarà più un luogo dove trovano...

probabilmente del cuore di questa riforma, perché si stabilisce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. L'emendamento che ho presentato in realtà - va riconosciuto il merito il merito - è stato presentato a nome di quattro associazioni di studiosi e di costituzionalisti, che si chiamano "Io Cambio", "Libertà Eguale", "Fondazione Magna Carta" e "Riformismo e Libertà".

Non sono tanto tranquillo, ma, insomma, mi fido di lei e ho piacere di avere dei Ministri *multitasking*. Dicevo che sono quattro associazioni importanti di studiosi e di costituzionalisti, che hanno avuto, rispetto a questa riforma, un approccio assolutamente aperto. Non si sono arroccati e rappresentano quella parte di società civile e di esperti che ritengono che sia importante pervenire a una riforma della nostra Costituzione e che sia importante fare in modo che questo meccanismo istituzionale così complesso, così circonvoluto e così farraginoso possa tornare a correre. Quindi hanno anche aperto alla possibilità che si arrivi a una soluzione Devo dire che, in modo apprezzabile, hanno messo a disposizione le loro competenze per fare in modo che alcune evidenti lacune del testo, soprattutto lacune di tipo tecnico, che pongono una sfida nell'applicazione

nel testo della Costituzione, così come è stato riscritto. Quando diciamo che il Governo è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni, in realtà diciamo tutto e non diciamo niente. Cosa significa che il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto? Significa, per esempio, che sarà Presidente del Consiglio la persona che prende anche un solo voto più degli altri? questo come si aggancia con la possibilità che il voto all'estero diventi decisivo? Noi abbiamo più di 5 milioni di elettori all'estero, che oggi sono sottorappresentati, perché per

Seconda domanda: il Presidente del Consiglio sarà il Presidente del Consiglio della maggioranza degli italiani oppure sarà semplicemente quello che prende un voto più degli altri, per cui, se ci saranno tre o quattro candidati, si potrà avere il premio di maggioranza con il 33-34 per cento dei voti? per cento dei voti? E poi cosa succede? Ci sarà un ballottaggio, forse? E cosa succede se, essendo le Camere ancora due ed essendo i voti separati, per qualche motivo dovesse esserci una distinzione o una differenza tra il risultato del Senato e il risultato della Camera? A quel punto, per esempio, ci sarebbe un ballottaggio? Su tutte queste questioni la maggioranza e il Governo non ci danno un testo che le chiarisce. votiamo un po' alla cieca, sostanzialmente, nel senso che ci fidiamo. Se votiamo sì, lasciamo un testo aperto di cui non sappiamo l'esito, anche perché la maggioranza non ha una posizione comune sulla legge elettorale che andremo ad adottare. Allora che cosa succede con questo emendamento? Questi studiosi e questi professori, tra cui ricordo il professor Ceccanti e Peppino Calderisi, hanno provato a identificare delle soluzioni.

di ritirarlo, perché desidero proteggerlo al fine della discussione che si terrà alla Camera.

e se stessimo facendo questa discussione sulla riforma costituzionale non così come abbiamo cominciato in queste settimane, con una serie di forzature da parte della maggioranza, con il contingentamento dei tempi, con l'assoluta indisponibilità di trovare un qualche terreno di confronto comune, reciproco, se fossimo per l'appunto in un altro clima, siccome tra l'ultima discussione che abbiamo fatto sul premierato e questa,

che hanno un carattere nazionale (elezioni europee naturalmente, non elezioni politiche, quindi non semplicemente elezioni regionali o comunali), abbiamo assistito al fatto che la maggioranza assoluta degli italiani non è andata a votare. Non era mai successo prima: 49,7 Siamo stati capaci di scendere sotto la soglia del 50 per cento degli aventi diritto. Non era mai accaduto, è la prima volta nel corso della storia democratica. Peraltro - lo sappiamo perché tutti quanti noi abbiamo letto i dati sull'astensione nelle ore immediatamente successive alla chiusura dei seggi - abbiamo riscontrato che nel giro di quindici anni si sono persi 10 milioni di elettori che non vanno più a votare, che guardano ormai alla politica come una cosa completamente separata. Peraltro, questa percentuale del 49,7 - come sappiamo e come abbiamo visto - da Roma in giù raggiunge dei livelli e dei numeri nettamente più alti. Nella mia città, che è la più grande del Mezzogiorno d'Italia, ha votato poco più di un cittadino su tre: questa è la condizione del nostro Paese. Ci darete atto, perché lo stiamo dicendo da molte settimane a questa parte, che questa dovrebbe essere l'unica grande discussione che facciamo. *(Applausi)*. Cosa si fa in un Paese in cui metà della popolazione non va più a votare? Si fa finta che questo problema non esista?

che sono, da molti decenni a questa parte, imperniate sul bipartitismo e nelle quali - come sappiamo - l'astensione è molto alta? Quindi, in qualche modo si minimizza questo dato e si crede che sia figlio semplicemente di una crisi democratica e non anche di tutte quelle motivazioni che hanno determinato e comunque hanno accentuato la crisi democratica stessa, oppure si prova a prendere di petto la questione?

l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'elezione del Parlamento per trascinamento, l'elezione diretta senza contrappesi, come sappiamo; insomma, le cose che stiamo ripetendo da molte settimane a questa parte. Ministro - che, rispetto a tale dato drammatico che attraversa la democrazia italiana in questa fase storica, questa che presentate sia effettivamente una riforma che produrrà degli effetti positivi? Penso che noi dovremmo discutere solo ed esclusivamente di questo. Questa riforma migliorerà la partecipazione democratica, oppure, nell'accentramento dei poteri che sottintende, renderà ancora più faticosa la partecipazione dei cittadini al gioco democratico e in qualche modo li escluderà da una dinamica dialettica che dovremmo invece provare faticosamente a ricostruire? Vorrei discutere di questo e i colleghi della 1a Commissione me ne daranno atto, perché nel corso di tutte queste settimane

della Repubblica italiana, che non esistono le scorciatoie; che le scorciatoie inevitabilmente ci metteranno in una condizione ancora più faticosa. Fermiamo questa discussione muro contro muro e cerchiamo di capire insieme quali possono essere i rimedi da mettere in campo. Penso che se si andrà avanti in questo modo, semplicemente con le forzature, il contingentamento dei tempi, le riforme costituzionali decise soltanto da una parte del Parlamento a scapito dell'altra, questi elementi di crisi sistemica saranno destinati ad allargarsi ancora di più e a metterci in una difficoltà sempre maggiore.

l'articolo 5 è un po' il cuore di questa riforma ed è l'articolo che introduce un *unicum* tra le democrazie occidentali, cioè l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. inoltre l'inserimento di un premio di maggioranza da tracciare con la legge elettorale in combinato disposto con l'articolo 6, prevede un altro *unicum*, ossia un Senato che rimane eletto su base regionale, tenendo conto però del premio di maggioranza nazionale. È come ghiaccio bollente, è un ossimoro:

fate quel passaggio che avete in animo e che è parte della vostra proposta agli elettori; proponete a quest'Aula di discutere qualcosa che abbia un senso: proponete qualcosa che noi non condividiamo comunque, ma che abbia un senso, ossia l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, perché quella è la vostra riforma. Fate questa proposta alle Assemblee del Parlamento e lasciate perdere questo abominio che è stato creato, che non ha né capo né coda, che stravolge i pesi e i contrappesi della Costituzione, che crea un *unicum*, che crea una decadenza di fatto del Parlamento. Tale riforma crea l'elezione di 600 figuranti che saranno appesi al Presidente del Consiglio e crea una stortura democratica e repubblicana che non ha pari in Europa. Lasciate perdere questo disegno proponete una cosa chiara. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica è nel vostro programma. I cittadini vi stanno dando fiducia: è evidente, l'abbiamo riconosciuto tutti. Questa maggioranza e questo Governo escono rafforzati dal voto europeo. europeo. Applicate il programma elettorale con cui vi siete presentati e facciamo una discussione seria sul presidenzialismo e sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Perché non lo volete fare? Perché proporre qualcosa che sconquassa completamente gli equilibri costituzionali? Ci troveremo di fronte a un Presidente del Consiglio pigliatutto, che ha l'investitura popolare, che ha una maggioranza che lo deve supportare per non tornarsene a casa, che potrà eleggere parte del o dei CSM, che deciderà, attraverso il Parlamento, quali sono i reati per i quali sarà ancora prevista l'obbligatorietà dell'azione penale, perché quello sarà un altro passo. Io credo sia più logico chiudere questa parentesi. Approviamo l'emendamento abrogativo del premierato ed iniziamo un ragionamento nuovo. Noi siamo contrari a uno stravolgimento costituzionale, anche in vista di un presidenzialismo reale, ma almeno avrebbe un senso: un senso di diritto costituzionale, un senso politico, un senso di mantenimento di una Costituzione che sta in piedi. Questo obbrobrio non sta in piedi e chiediamo a maggioranza e Governo, che si sono visti confermata la fiducia da parte del Paese, di fermarsi e di fare invece una cosa sensata.

Signor Presidente, stiamo illustrando le proposte emendative delle opposizioni a questo articolo 5. Come è stato detto in precedenza, dal nostro presidente Patuanelli, esso è il cuore di questa riforma, quello che attribuisce un premio di maggioranza e che stabilisce la durata del mandato del *Premier* eletto.

con cui questa riforma è stata scritta e sottoposta alla Commissione è indice e spia dell'approccio raffazzonato e frettoloso con cui questa maggioranza si è approcciata ad una materia tanto delicata. Dico questo perché nella prima versione, che poi è stata emendata dallo stesso Governo di fronte alle nostre rimostranze, si diceva del *Premier* eletto che aveva una durata soltanto di cinque anni, senza dire nulla su quanti mandati potesse ricoprire, dando quindi per implicito che, non essendoci un termine, poteva ricoprirne *ad libitum*, in eterno. Quindi, un *Premier* eletto che poteva essere potenzialmente rieletto per sempre. Un abominio, una cosa assolutamente spaventosa: quindi, vi siete auto corretti e avete detto che, sì, può restare in carica per due legislature al massimo, ma in realtà sono due legislature e mezzo, se non arriva a completare la metà quindi, dando un *escamotage*. Neanche questo, però, è sufficiente, perché un *Premier* che ha in mano il Parlamento e che ne detiene il potere di vita o di morte può presentare delle dimissioni pretestuose, delle dimissioni che siano minacciose verso il Parlamento e costringere il Parlamento successivo a riconfigurarsi in base ai propri desiderata. Voi capite bene che questo, con la democrazia, non ha nulla a che vedere. Qui si viene al secondo punto, che io trovo particolarmente spaventoso e che è spia o di profonda ignoranza o di profondissima malafede. Da parte di prominenti esponenti di questa maggioranza, si è colta l'occasione di quanto è accaduto in Francia a seguito delle elezioni europee, ossia dello scioglimento da

o mentite in malafede o siete profondamente ignoranti, perché quello che è accaduto in Francia è l'esatto contrario: il presidente Macron rimarrà lì anche qualora le elezioni che egli ha indetto a fine giugno dovessero stabilire una maggioranza all'interno dell'Assemblea nazionale di colore completamente diverso dal suo. Questo non ha nulla a che fare con quello che state facendo voi, che invece disegnate un Parlamento, quindi la sede della rappresentanza popolare, dei rappresentanti del popolo completamente asservito ad una sola persona, un Parlamento come è stato detto in precedenza. È davvero scandaloso, quindi, che vogliate provare a far passare il messaggio di dare più potere al corpo elettorale quando gliene togliete; come è stato detto, della legge elettorale non c'è traccia, quindi non si sa con quale tipo di legge elettorale volete poi implementare questa riforma che scivola davvero verso il potere assoluto messo nelle mani di una sola persona. Davvero non è possibile tollerare una simile menzogna. Dite quantomeno la verità agli italiani: questo sistema non ha nulla a che fare con il sistema francese. È un sistema che vi siete inventati voi *in vitro* e che non porterà nulla di buono al Paese.

dovrei soffermarmi ad illustrare gli emendamenti a mia prima firma che sono un tentativo subordinato di rimediare a una riforma che ha degli elementi che ci fanno capire che non c'è nulla di irimediabile

come abbiamo sottoscritto altri emendamenti soppressivi di articoli di questa riforma. Sono convinto che anche la maggioranza si sia resa conto che questa riforma è partita male, che sono stati fatti dei rattoppi anche da parte della stessa maggioranza, perché ha capito che la riforma era nata male. È una riforma che tradisce gli elettori, nella misura in cui si è data, in campagna elettorale, l'illusione che si volesse rafforzare il Presidente della Repubblica e poi si è cambiata rotta e si è inserita questa ipotesi del premierato, su cui neppure si dice la verità, perché ancora oggi si sta continuando a dire che si tratta solo di elezione diretta, di cui parla questo articolo, ma ci sono altre norme che invece scardinano la nostra Costituzione. Signor Presidente, per suo tramite vorrei fare un appello a quei colleghi della maggioranza che sono dei giuristi non per titolo conseguito, quindi non perché sono avvocati, ma perché hanno cultura giuridica, perché amano i princìpi generali del diritto, perché amano la giustizia e perché sono innamorati della Costituzione perché sanno che è stata costruita come se fosse un'opera d'arte. Posso capire che, per esigenze di coesione nella maggioranza, daranno il loro voto per portare avanti questa riforma, ma li inviterei almeno ad aprire una riflessione e un confronto all'interno della maggioranza stessa. Sono infatti convinto che altrimenti dovremmo veramente preoccuparci se c'è una voce unica e univoca anche all'interno, se non c'è un dibattito interno che mette in discussione quella che si sta presentando come una riforma dilettantistica del diritto costituzionale, come un obbrobrio di diritto costituzionale. Se consideriamo la Costituzione come se fosse un'opera d'arte, non è che non si possa intervenire: andiamo da un restauratore se vogliamo restaurare un dipinto di Monet. Se però restauriamo un dipinto di Monet deve uscir fuori un dipinto di Monet: può bastare una pennellata, un ritocco per correggere qualche minimo errore che il tempo magari gli ha consegnato. smantellando i princìpi cardine della Costituzione. È come se su quel quadro di Monet ci fosse una macchia di sugo: il quadro non ha più il suo valore. Voi state scardinando gli elementi del diritto, per questo mi rivolgo ai giuristi: come fate a concepire una democrazia in cui non si rispetta lo Stato di diritto e quel bilanciamento tra i poteri che i Padri costituenti hanno inserito proprio per garantire la la democrazia? Senza il bilanciamento dei poteri non c'è democrazia, c'è autoritarismo, c'è il pericolo da cui proprio i Padri costituenti volevano metterci in guardia.

darci una risposta: come ritiene, signora Ministro, che questa riforma sia compatibile con lo Stato di diritto, con il bilanciamento dei poteri e con la democrazia? Per favore, ce lo dica.

farò precedere la mia valutazione di merito da una richiesta sull'ordine dei lavori, perché, se non ho calcolato male i tempi, con questo intervento dovrei esaurire il tempo assegnato al Gruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe. Pertanto, signora Presidente, essendo noi a pagina 149 del fascicolo dovendo arrivare fino a pagina 519, le anticipo sin d'ora la richiesta formale da parte del nostro Gruppo di un'estensione dei tempi al fine di poterci consentire di entrare nel merito delle discussioni dei successivi emendamenti, tenuto conto del fatto che, come abbiamo più volte detto, l'atteggiamento e l'impostazione del nostro lavoro è stata tutt'altro che

che venga acquisito agli atti e che poi la Presidenza ne tenga in debito conto e formuli una risposta che ci consenta di intervenire. Passando invece alla questione essenziale dell'articolo 5, già altri colleghi hanno fatto una serie di rilievi, ma questo articolo rimanda, dal nostro punto di vista, alla bontà dell'ordine del giorno che avevamo presentato e che con eccessiva superficialità il Governo e il relatore hanno chiesto all'Assemblea di respingere. Noi avevamo chiesto che l'esame completo del provvedimento venisse subordinato alla necessaria

il meccanismo elettorale. Come è noto, in sede di Assemblea costituente si discusse molto se costituzionalizzare o no il meccanismo elettorale che allora vigeva, che era il sistema proporzionale, e, attraverso una valutazione fatta dai nostri Padri costituenti, si decise di non irrigidire la Carta costituzionale con il meccanismo della legge elettorale. Questo consentì alla nostra Repubblica di affrontare il passaggio e la crisi alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta, con l'introduzione di una nuova legge legge elettorale con un sistema maggioritario. Tale sistema consentì da quel momento la formulazione di una diversa modalità con la quale il sistema politico si reggeva e si orientava. Ora noi andiamo ad introdurre questo elemento in maniera fissa e rigida all'interno della nostra Carta costituzionale. Addirittura originariamente vi era una previsione di un numero sancito, il 55 per cento di premio di maggioranza, senza peraltro immaginare quale fosse la soglia minima affinché questo consentisse un equilibrio, cosa che peraltro è già prevista perché vi è già un monito esplicito da parte della Corte costituzionale all'interno della valutazione fatta nella legge del cosiddetto Porcellum. per cento è stato poi tolto, ma permane l'elemento del premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere. E qui viene a galla il nodo; nodo; noi manteniamo inalterati l'articolo 56, che stabilisce che la Camera dei deputati viene eletta su base nazionale, e l'articolo 57, che stabilisce che il Senato della Repubblica viene eletto su base regionale, e poi diciamo che bisognerà introdurre un premio di maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Voi capite che questo elemento inevitabilmente ci porta a dover chiedere come questo si farà. Se infatti noi facciamo un'operazione di questo genere prima di avere chiarito come questo meccanismo arriverà a terra, potremo trovarci in una duplice condizione: quella di non avere una legge elettorale alla fine di questo provvedimento, perché non c'è scritto da nessuna parte che si potrà approvare una legge elettorale prima che questa norma diventi operativa, quella di avere una legge elettorale che confligga con questa previsione. Quindi, signora Presidente, diventa indispensabile bloccare l'articolo 5, aprendo prima una discussione reale sul contenuto politico della legge elettorale. Diversamente noi trasferiamo alla Camera

e ammettiamo che questo testo non può stare in piedi dal punto di vista degli equilibri costituzionali.

Grazie.

disegno di legge. Vi abbiamo chiesto a più riprese di fare questa discussione aprendo il confronto, pensando che stiamo maneggiando - e lo dobbiamo necessariamente fare con cautela la Carta costituzionale che ha tenuto in piedi la nostra Repubblica in questi anni. Voi l'avete voluto politicizzare, ne avete voluto fare - come abbiamo detto - oggetto di scambio per la tenuta della maggioranza e lo avete voluto fare, ovviamente, a ridosso di un'importante tornata elettorale. A me in questo momento verrebbe difficile non chiedervi almeno di essere coerenti con una scelta che noi vi abbiamo scongiurato di non fare: ignorare, da questo punto di vista, che anche in un quadro di oggettiva tenuta del risultato elettorale del risultato elettorale però qualche messaggio chiaro viene. In questo intervento, illustrando le ragioni di questo emendamento, che chiede sostanzialmente di cancellare questa norma, due passaggi. Il primo riguarda il voto nel Mezzogiorno d'Italia, che - è evidente - vi dà un chiaro campanello d'allarme su una delle riforme oggetto di questo scambio, una delle principali, uno dei pilastri, uno dei piedi di queste riforme. Il Sud chiaramente vi dice: fermatevi sull'autonomia, fermatevi su questo scambio che state giocando sulla pelle del Paese e che state facendo sostanzialmente per tenere in piedi il vostro equilibrio. Questa riforma oggi è un pezzo di questo ragionamento; ignorare quell'esito e quella voce così chiara così netta sarebbe, secondo noi, un vostro ulteriore segnale di incoerenza. Venendo però al merito, è vero che questo articolo è esattamente il cuore. Vorrei proprio prendere il testo per capire. Ci avete ripetuto a più riprese, ci avete detto e ridetto che non toccate i poteri del Presidente della Repubblica. Ma con semplicità, visto che si tocca l'articolo 92, il Presidente della Repubblica - così recita la nostra Carta costituzionale al secondo comma comma dell'articolo 92 - «nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri». Così come lo riformulate adesso, «Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto»; poi, scendendo giù, «Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo». Mi sembra così chiaro che non sarebbero necessari commenti. In un caso è il Presidente della Repubblica che nomina il Presidente del Consiglio; in un altro caso, nel vostro testo, conferisce un incarico al Presidente eletto.

Fate riferimento alla rappresentatività, sotto nostra sollecitazione, ma, in ogni caso, il pilastro di questa norma è che il Presidente della Repubblica deve sostanzialmente prendere atto della scelta degli elettori. Voi dite: ma noi facciamo scegliere a suffragio universale e diretto, quale prova più democratica? Noi abbiamo provato a spiegarvi, e continuiamo a farlo in questo passaggio, che questa non è necessariamente di per sé una prova di democrazia. Anzi, questa prova

si cancellano gli equilibri costruiti dai nostri Padri e dalle nostre Madri costituenti e soprattutto si cancella la centralità del Parlamento stesso, che è l'unica voce che diamo ai nostri cittadini nel momento in cui gli chiediamo di scegliere. Il Parlamento in questo caso non conterà e non si esprimerà più attraverso l'istituto della fiducia, che vedremo poi, nel corso degli articoli che verranno, cambiato radicalmente nel suo essere, mentre il Presidente della Repubblica dovrà conferire un incarico prendendo atto di quella che è la volontà degli elettori. In tal senso, in questo articolo si fa anche riferimento a un altro passaggio. Anche qui ci potrebbe essere qualche contraddizione: nomina e revoca. Qualcuno ci ha detto, nel dibattito in Commissione: ma come, avete sempre chiesto che alla nomina fosse abbinata la revoca. E noi abbiamo provato così a spiegarvi: attenzione, nomina e revoca, in un contesto nel quale

quanto scelto dal Parlamento. Un ultimo passaggio e chiudo. In questo articolo voi fate riferimento alla legge elettorale. Il senatore De Cristofaro ha fatto chiaramente riferimento alla scarsa partecipazione anche in questa tornata elettorale, che dovrebbe essere un assillo per tutti noi. Noi vi abbiamo più volte ribadito che una legge elettorale, per quanto riscritta e quindi passando dal 55 per cento - così come lo recitate qua - a un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere, detto così, senza definire una soglia sulla base sulla base della quale scatterebbe questo premio, non solo viola le norme e gli orientamenti varati dalla nostra Corte costituzionale, ma è un *vulnus* pesante alla nostra democrazia, di fronte al fatto che, insieme a sempre più scarsa partecipazione, c'è una grande frammentazione del quadro politico. Quindi, noi ci troveremo di fronte alla possibilità che tutto - Parlamento, *Premier* e tutti gli organi di garanzia eletti dal Parlamento - sarebbe nelle mani di una maggioranza che è espressione di una minoranza di di un'ulteriore minoranza: un *vulnus* democratico inaccettabile che noi stiamo provando a evidenziarvi in questo dibattito, per quanto molto vi mostriate sordi e assolutamente indifferenti, in spregio a quello che è lo spirito vero che ha ispirato la nostra Costituzione e che allora ha ispirato i nostri Padri e Madri costituenti.

a richiamare, anche in relazione all'ultimo dato elettorale che c'è stato qualche giorno fa, quello che è accaduto nel Mezzogiorno d'Italia: la scarsissima partecipazione al voto e il possibile, anzi probabile collegamento tra questo evento e il dibattito sull'autonomia differenziata, che certamente non aiuta e non mette il Sud in quella condizione che meriterebbe. Come sappiamo, quello è un provvedimento, per quanto non sia una riforma propriamente

evidentemente di porre in luce quali sono le storture, almeno secondo noi, di quello che consideriamo l'articolo più pericoloso e sbagliato, quello che prevede l'elezione diretta, a suffragio universale, del Presidente del Consiglio per cinque anni; cinque anni che però, ricordiamolo, possono diventare dodici anni e mezzo, causando, naturalmente, in questo modo una vera e propria trasformazione radicale della scelta di governo, per di più con un argomento puramente propagandistico. Quando faremo il *referendum* confermativo ci sfideremo su questo punto e cercheremo di dimostrare com'è falsa questa narrazione, quella secondo cui questa riforma costituzionale darebbe ai cittadini la facoltà di scegliere il Presidente del Consiglio. Come sappiamo perfettamente, questo è davvero un artificio retorico, perché per consentire ai cittadini di un Paese, nella fattispecie del nostro Paese, di scegliere il Presidente del Consiglio, non serve una riforma costituzionale come questa. Questa riforma costituzionale serve non a scegliere il Presidente del Consiglio, ma a dare al Presidente del Consiglio molti più poteri di quelli che ha oggi e, soprattutto, serve a limitare in maniera molto significativa Se il tema fosse semplicemente la scelta del Presidente del Consiglio, quindi dare alla popolazione la facoltà di esprimersi effettivamente su questo, basterebbero degli accorgimenti molto più semplici. Basterebbe, per esempio, una legge elettorale diversa da quella con cui andiamo a votare da molti anni a questa parte, oppure basterebbero alcuni accorgimenti costituzionali, come quelli che esistono nel modello tedesco. Lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo presentato degli emendamenti che vanno in questa direzione, prendendo a riferimento un modello, come quello che si usa in Germania, che cerca di salvaguardare o comunque di tenere assieme quelli che dovrebbero essere i due elementi di fondo utili allo sviluppo di un percorso democratico in una democrazia: la stabilità di governo, che certamente è un valore e ha un elemento di un elemento di densità attorno alla quale fare un ragionamento, e il tema della rappresentanza, che invece - come sappiamo - in questa proposta di riforma che arriva dai partiti di centrodestra viene completamente abbandonato al suo destino. accentrare i poteri nelle mani di una sola figura come quella del Presidente del Consiglio eletto dal popolo e determinare l'elezione del Parlamento per trascinamento significherà inevitabilmente ridurre in maniera molto significativa la rappresentatività così come l'abbiamo conosciuta.

Credo che in questo caso anche la maggioranza dovrebbe votare questo emendamento soppressivo per un dovere di onestà nei confronti dei vostri elettori. Mi perdoni, Presidente, ma mi rivolgo alla maggioranza tramite lei. Dovreste votarlo perché in campagna elettorale avete detto che avreste rafforzato i poteri del Presidente della Repubblica; che si trattava di una forma di partecipazione dei cittadini per eleggere il Presidente della Repubblica. Allora per un dovere di onestà o cancellate questa norma o la riscrivete togliendo le parole «Presidente del Consiglio» e scrivendo le parole «Presidente della Repubblica», anche se poi dovreste cancellare anche tutti gli altri articoli. C'è un dovere di onestà anche nei confronti dei cittadini che state continuando a illudere. Ho visto un video della Meloni in cui parlava del premierato e faceva vedere le immagini di tutti i Presidenti del Consiglio, dicendo che sono tutti frutto di opere del Palazzo. molto bello il video, ma non diceva la verità, poiché manca tutta la seconda parte della riforma, che smantella la Costituzione, marginalizza il Parlamento, toglie poteri al Presidente della Repubblica e crea l'immagine di un *Premier* assoluto,

l'autoritarismo, quando cercano l'uomo forte, normalmente questo succede in momenti di crisi, di paura, di difficoltà, quando i cittadini devono affrontare dei demoni interni e non riescono a farlo, quindi vogliono il salvatore. Io penso che gli italiani non abbiano bisogno del salvatore. Dite loro come stanno le cose. Il mio è un appello ad essere intellettualmente onesti. Finitela con questa storia dell'elezione diretta, perché l'elezione diretta è soltanto una parte di questa riforma, è soltanto l'inizio di un comma dell'articolo 5 e basta, poiché il resto è lo smantellamento dei principi costituzionali che ci difendono dall'autoritarismo. Se le persone vogliono loro autoritarismo, dobbiamo chiederci anche altre ragioni: perché vogliono l'autoritarismo? Spesso questo desiderio nasce perché ci si illude che il *leader* possa dare delle soluzioni semplici a problemi che sono complessi e tutti voi sapete che sono complessi. È semplice parlare di promesse irrealizzabili: la *flat tax*, abbassiamo le tasse tutte al 20 Poi c'è un bagno di realtà quando si sta al Governo, come un bagno di realtà ha fatto la Meloni quando faceva quello *sketch* comico e parlava delle accise sulla benzina

Non so se tutti i cittadini hanno visto le due versioni della Meloni nello *sketch* e della Meloni presidente del Consiglio. Ci si consegna all'illusione che la realtà complessa si possa risolvere con il *leader* che fa le cose semplici, o meglio con il semplicismo, perché poi è facile parlare di immigrazione e dire «facciamo il blocco navale», che poi di fatto non si fa. Poi bisogna cominciare a rendersi conto che invece c'è bisogno di affrontare il problema anche alla radice e che c'è bisogno di cooperazione internazionale.

Signor Presidente, questo emendamento è esemplificativo della nostra posizione per quanto riguarda la necessità di apportare miglioramenti alla nostra forma di governo parlamentare. Non siamo semplici difensori dello *status quo*,

un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, che, contrariamente a quanto fa credere la maggioranza con il suo progetto, possono essere potenziati in maniera ragionevole, non irragionevole, senza per forza dissestare e gli equilibri costituzionali e farci uscire dalla forma di governo parlamentare con trovate ingegnose, ma molto, molto rischiose per la tenuta del nostro ordinamento e per la qualità stessa Com'è noto, nelle nostre proposte ci ispiriamo agli elementi qualificanti del modello di governo tedesco e della forma di governo tedesca, che è una forma di governo parlamentare razionalizzata, in quanto concilia la salvaguardia dell'autorevolezza del Parlamento, che invece la vostra riforma distrugge e cancella, con una stabilità dei Governi, che a più riprese ha dimostrato di essere molto, molto forte. Il segreto di questa forma di governo è di porsi problemi di funzionamento delle istituzioni senza far saltare gli equilibri che esistono tra i principali poteri dello Stato (il Primo Ministro, da una parte, il Parlamento, dall'altra, e il Presidente della Repubblica, da un'altra ancora). Contrariamente a quanto molti hanno sostenuto anche in questo dibattito, non è affatto vero che la figura del Presidente della Repubblica da un sistema siffatto viene svuotata o ridotta ad una funzione cerimoniale. Non è affatto così, come dimostra la storia dei Paesi in cui questa forma di Governo è stata applicata. Su tutte le questioni fondamentali (dalla nomina della persona da inviare alla Camera politica per ottenere la fiducia dei deputati, dove il sistema ha una sola Camera che vota la fiducia, fino alla procedura di eventuale scioglimento anticipato delle Camere), il Presidente della Repubblica, in un sistema siffatto, che comprende la sfiducia costruttiva e altri punti che con i nostri emendamenti abbiamo proposto, mantiene la possibilità di incidere sulle scelte fondamentali dell'indirizzo del Paese in un momento di emergenza, possibilità che perde del tutto con lo sgangherato sistema che il disegno di legge n. prefigura e che, sostanzialmente, come hanno ben spiegato anche molti colleghi nello scorcio di dibattito che c'è stato quest'oggi, si traduce in un immotivato e irragionevole trasferimento di una quantità abnorme di potere nelle mani del Capo del Governo, il quale, complice il premio di maggioranza, si trova a disporre insieme della vita del Parlamento, della elezione del Presidente della Repubblica e della possibilità di nominare la maggioranza dei membri della Corte costituzionale: direttamente, infatti, lo fa un Parlamento che che è sotto il suo controllo per cinque unità; indirettamente, lo fa un Presidente della Repubblica, che è sotto il suo controllo, per le ragioni che abbiamo detto, che ne nomina altri cinque. Questo disprezzo per i contrappesi, questa concentrazione del potere senza compensazioni e senza riguardo alla sorte degli altri organi costituzionali è molto pericolosa va in direzione opposta rispetto al progetto di miglioramento istituzionale che invece noi cerchiamo di proporre con emendamenti come questi, che sono i nostri più qualificanti e che, non a caso, sono stati firmati dal nostro capogruppo Boccia. Quindi, nel dichiarare il voto favorevole a questo emendamento, noi facciamo anche un ulteriore appello alla maggioranza, affinché smetta di usare parole ingannevoli su quali siano gli intendimenti di fondo del suo del suo progetto. Se, infatti, l'intendimento di fondo è aumentare la stabilità e l'efficienza dei Governi, lo si può fare senza portare lo scompiglio nella nostra Costituzione. Evidentemente, non è quello l'obiettivo. Non avete l'obiettivo di aumentare la stabilità e l'efficienza dei Governi; avete l'obiettivo di realizzare una concentrazione eccessiva del potere. Tra l'altro, ho sentito in questi giorni qualcuno sostenere: l'affluenza è bassa? La risposta è il premierato. Peccato che l'affluenza sia stata bassissima in elezioni amministrative, dove c'è l'elezione diretta del capo dell'amministrazione. Anche questa affermazione, dunque, è stata un modo di arieggiare il sistema respiratorio, ma non si è avvicinata molto alla realtà dei fatti.

puramente ostruzionisti, perché ho sempre sostenuto che, quando c'è in ballo il destino della nostra Costituzione, è tutto lecito, compresi, naturalmente, gli emendamenti ostruzionistici. Tra quegli emendamenti, però, ve ne erano anche tanti di merito.

più che al tema della stabilità, riconosco che esiste nel nostro Paese obiettivamente un problema che riguarda anche la stabilità. Riconosco che ci sono stati negli anni troppi Governi e quando viene snocciolato il numero molto significativo di Governi che nel corso degli anni si sono avvicendati in Italia e in qualche modo questo viene richiamato come un significativo problema politico, ammetto che questo problema esiste, lo vedo, lo considero effettivamente un tema attorno al quale provare a costruire un ragionamento, ma sono convinto che se il problema fosse stato questo, cioè dare all'Esecutivo maggiore stabilità, si sarebbero potute ricercare delle soluzioni - una per tutte, l'abbiamo ripetuto fino a sgolarci: la sfiducia costruttiva - che non prevedevano questo clamoroso stravolgimento costituzionale, che probabilmente da quest'Aula parlamentare sarebbero state votate all'unanimità o comunque a larghissima maggioranza e che avrebbero cercato di costituire contemporaneamente un elemento di salvaguardia al tema della stabilità, senza però intervenire in maniera così così dirompente sul tema della rappresentanza. Si è scelta, invece, un'altra strada, peraltro a colpi di maggioranza, quindi rinunciando a un minimo elemento di dialogo. Indiremo il *referendum*, come è noto, perché arriveremo con due proposte purtroppo incompatibili e inconciliabili. Fortunatamente, la saggezza dei Padri costituenti tanti anni fa aveva previsto che, nel caso in cui non ci fosse stata la maggioranza dei due terzi in Parlamento, si sarebbe concluso il percorso della riforma costituzionale dando la parola al popolo sovrano ed effettivamente questo succederà. Considero anche questo *iter*, francamente, in una fase come questa, di crisi così seria della democrazia del nostro Paese, purtroppo una forzatura e lo considero un'operazione clamorosamente propagandistica. Non è vero che si sta dando ai cittadini italiani la facoltà e la possibilità di scegliere il proprio Presidente del Consiglio, perché questo avviene già oggi: ma davvero c'è qualche cittadino italiano che, quando ha votato un anno e mezzo fa alle elezioni politiche, non sapeva che dando la maggioranza a Fratelli d'Italia, alla Lega e a Forza Italia sarebbe diventata presidente del Consiglio

i partiti di destra un anno e mezzo fa sceglievano quale Presidente del Consiglio immaginare e da chi farsi rappresentare. Quindi, quel diritto di scelta, come si vede, esisteva già. In questo caso, non stiamo parlando del diritto di scelta, di scelta, ma dei poteri e delle prerogative, che sono una cosa totalmente diversa dal diritto di scelta e stiamo parlando del rischio molto grave che questa concentrazione di poteri avvenga sulla pelle del pluralismo. Questo è il punto che non quadra di questo ragionamento. Mi dispiace anche che i colleghi di centrodestra non parlino mai e non si confrontino rispetto ai temi che stiamo sollevando, ma mi pare che questi siano gli aspetti di gran lunga più significativi della riforma.

potremmo conoscere prima come si intende applicare il canguro, giusto per poter organizzare gli interventi? Abbiamo preso atto, ma non ci siamo rassegnati a un dibattito sulla riforma costituzionale che vede applicati sia il canguro sia il contingentamento dei tempi, signora Presidente. Non ci rassegniamo, almeno diteci con quale criterio applicate questi due istituti!

farò da tramite nel riproporla e facendo conoscere al Presidente questa richiesta, su cui però ho l'obbligo di dire che nelle precedenti Conferenze dei Capigruppo la Presidenza si è già pronunciata.

lei ha detto, i temi sono salienti. Converrà con me che condensare in un minuto la possibilità di intervenire a questo punto 350 pagine di fascicolo è praticamente impossibile, quindi al momento prendo atto del fatto che noi abbiamo esaurito il nostro tempo e che, allo stato, non ci è data la possibilità di intervenire ulteriormente. Chiedo che questo venga messo a verbale per tutte le considerazioni successive, perché significa che non siamo neppure alla metà dell'esame parlamentare della riforma della Costituzione e un Gruppo dell'opposizione non ha più la possibilità di intervenire nel merito.

non hanno sufficienti poteri e quindi c'è bisogno di rafforzarli. È una palese menzogna in quanto già in questa legislatura si può vedere come il Governo stia governando senza incontrare alcun tipo di ostacolo sulla propria strada. Ho avuto già modo di ricordare che da quando

potendo egli proporre la propria squadra di Ministri al Presidente della Repubblica, che ha poi il compito di investirli del ruolo e del potere di Ministri, non ha

che non stravolgerebbe tutto l'assetto del rapporto dei poteri, del potere esecutivo del Governo e del potere legislativo del Parlamento, così come invece fa questa riforma. Essa infatti non si limita a dire votare il Primo Ministro, ma fa uno scatafascio di tutto il resto, cosa di cui ovviamente la maggioranza si guarda bene dal

di buonsenso. Se un Ministro, per una qualunque ragione, non è più in grado di ricoprire quel ruolo, è chiaro che il Primo Ministro deve poterne proporre le dimissioni. Credo che un emendamento del genere possa soltanto incontrare il favore della maggioranza, che appunto lamenta lo scarso potere

che stanno forzatamente proponendo e che noi ovviamente non condividiamo minimamente. Continuo a dire e voglio denunciare in ogni sede che il fatto che sia stata messa una limitazione temporale alla possibilità, di discutere la riforma è assolutamente vergognoso e dimostra un approccio antidemocratico, proprio laddove invece dovrebbe essere il più democratico, il più aperto e di maggiore condivisione possibile, ossia nella modifica della nostra Carta costituzionale.

almeno introdurre una pausa, per consentire alla maggioranza di riflettere su quello che sta succedendo. Qui va soppressa l'elezione diretta del *Premier*, perché non si tratta di elezione diretta del *Premier*. Cambiate nome a questa figura istituzionale, perché non è la stessa: questo dovete dirlo ai cittadini, non è assolutamente il *Premier* inteso come la figura istituzionale che fino ad oggi rappresentava l'Esecutivo. Applaudo anch'io. È la stanchezza che a volte fa questi scherzi. Se noi eleggiamo una persona che ha potere di ricatto sul Parlamento, stiamo introducendo una distorsione del sistema democratico ed è una cosa gravissima. Voi dovete dirlo ai cittadini, perché questo i cittadini non lo sanno. State continuando a mentire sapendo di mentire. C'è un silenzio imbarazzante del Governo, che ancora non è stato in grado di rispondere a una domanda, che allora ripeto: che allora ripeto: come fate a pensare che questo sistema sia compatibile con lo Stato di diritto? Come fate a pensare che questo sistema sia compatibile con l'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea, dove lo Stato di diritto è è fondamentale, dove la divisione dei poteri è fondamentale e dove non si può parlare di democrazia senza la divisione dei poteri? A cosa servirà questo Parlamento? A cosa serviranno i parlamentari che dovrebbero essere i rappresentanti della popolazione? State dando uno schiaffo in faccia ai cittadini e direte che i loro rappresentanti non contano nulla. Lo avete già fatto, perché nel mio territorio, dove c'è il problema del sisma, avete un parlamentare della maggioranza, che è anche commissario al sisma, non vi siete accorti di averlo. Avevate fatto una prima stesura di un provvedimento sul superbonus che aveva bloccato la possibilità di ricostruire nelle aree terremotate. Ecco l'interesse che ha questo Governo nei confronti dei cittadini: rendere inutilizzabili e inutili i parlamentari. Questo lo state già facendo e lo volete istituzionalizzare. Questa figura perché la chiamate *Premier*? Avrà il potere legislativo. Avete respinto gli emendamenti che proponevano di modificare l'articolo 77 della Costituzione proprio per evitare l'usurpazione del potere legislativo da parte dell'Esecutivo. Quelle proposte volevano evitare che si potessero fare dei decreti legge laddove l'urgenza non c'è, o dei decreti *omnibus* con cui di fatto si sta facendo un'invasione di campo. Si marginalizza il Parlamento, che non fa altro che approvare e convalidare i vostri decreti e qualche spazio per i disegni di legge viene riservato a quelli di iniziativa governativa. Un'elezione diretta oggi è pericolosissima, signora Presidente, perché non abbiamo alcuno strumento per tutelare i cittadini dalla manipolazione, dai tentativi di manipolazione delle masse, dalle promesse elettorali fasulle, che si sanno essere fasulle. L'unica protezione che hanno i cittadini per la loro libertà e per la democrazia la dà la Costituzione e voi questa Costituzione la state smantellando.

il cosiddetto *Premier* eletto può mandare a casa quando vuole i parlamentari e se, quando viene eletto, trascina il Parlamento che è a lui collegato, davvero c'è un problema di democrazia

In questi giorni molti italiani sono contenti dei campionati europei. Voi invece negate, ad esempio, la fotografia del risultato dei campionati europei: è una dissociazione tra la realtà sociale del Paese e il modo in cui si vuole governarla. Da una parte applaudiamo e siamo tutti contenti che si vada in questa direzione, ma non ci accorgiamo che si tratta di una società multietnica

Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento perché siamo fortemente contrari, se ancora non si fosse capito, ai contenuti di questa riforma e in particolare alle norme previste dall'articolo 5, che prevedono anche un premio di maggioranza e l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Noi non siamo a favore di questa previsione. Riteniamo che non ci sia un bilanciamento dei poteri dello Stato. Noi riteniamo che non sia corretto derogare a quanto prevede la nostra Costituzione, che attribuisce questa prerogativa al Capo dello Stato, come abbiamo più volte ribadito anche durante le votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 1. Ritengo che, per quanto la maggioranza non faccia altro che dire che in questo modo noi conferiamo ai cittadini il diritto di scegliere chi li deve governare, dimentichiamo che la nostra Costituzione prevede una separazione tra il potere legislativo e quello esecutivo. In questo modo, con questo sistema elettorale, con le previsioni di questo articolo, noi cancelliamo completamente tale separazione, perché facciamo avvenire la scelta all'interno della stessa elezione elezione da parte dei cittadini. Tutti i Paesi che hanno un presidenzialismo, che però in quel caso è rivolto al Presidente della Repubblica, o comunque una elezione diretta del Capo del Governo hanno una separazione spaziale e temporale dell'elezione delle Camere e quindi del potere legislativo. Noi, invece, con questa fattispecie, all'interno di questo provvedimento, mettiamo insieme le due elezioni, facendo un minestrone, un *unicum* che non è presente in nessun'altra democrazia democrazia in tutto il globo terracqueo, per usare una immagine cara all'attuale *Premier*. Secondo noi, o separiamo le due elezioni oppure è meglio restare col sistema attuale. Per questo, ribadisco il voto a favore di questo emendamento.

ma dobbiamo anche renderci conto del contesto nel quale state costruendo questa elezione plebiscitaria: lo state facendo senza fissare delle regole che proteggano i cittadini, ma ci stiamo rendendo conto di quello che succede durante le campagne elettorali? Intanto, siete stati in qualche maniera protagonisti di una sorta di manipolazione, perché in campagna elettorale si è parlato di tutto: della *flat tax*, del blocco navale, di tante promesse elettorali che si sapevano irrealizzabili. Se non c'è un sistema che protegge i cittadini da questo, come potete pensare di costruire un sistema dove il potere nasce più che altro sulla sulla base di un applauso, dove non c'è più la votazione per le istituzioni? Non si voterà più per le istituzioni, ma si voterà per il mito per il mito dell'uomo forte, non si voterà più per il Parlamento perché sarà un voto a strascico, ma soprattutto a cosa servirà votare per un Parlamento che non potrà sfiduciare facilmente il *Premier*, il *Premier*, che sarà costantemente sotto ricatto, per un Parlamento che questo *Premier* da un giorno all'altro potrà decidere di mandare a casa senza motivi, discrezionalmente, come vuole? Lui si potrà dimettere e mandare tutti a casa. Immaginate il potere ricattatorio che potrà avere questo uomo forte. Voi state giocando su una sorta di regressione sociale. Succede sempre così: quando c'è la volontà dell'autoritarismo, dell'uomo forte al potere, c'è sempre alla base una crisi sociale, una crisi di identità, una crisi economica, una crisi di valori. I cittadini, in una condizione di fragilità, in una condizione sociale di paura, hanno bisogno del salvatore e voi volete proporre questo salvatore dimenticando quali sono i reali problemi della democrazia. Noi abbiamo un Parlamento che è costantemente umiliato da un Esecutivo che ha usurpato il potere legislativo. Di fatto è così, noi ce la raccontiamo e, invece di risolvere questo problema democratico, voi lo state peggiorando e non so quale immagine dell'Italia vorrete dare all'Europa e al mondo intero.

una giurisprudenza costituzionale per cambiare i principi fondamentali della Costituzione occorrerebbe un diverso orientamento del potere costituente e quindi una nuova Assemblea costituente. Un pasticcio che più si approfondisce e più rivela la grande presa in giro che contiene questa riforma, che parte da lontano, dalla vostra campagna elettorale, come abbiamo detto tante volte, ma lo ribadisco anch'io. In campagna elettorale non avete mai parlato di premierato, bensì di presidenzialismo, e nei giorni scorsi, davanti a questa ennesima osservazione, qualcuno dai banchi della maggioranza ha gridato qualcosa che sostanzialmente voleva dire dire che il premierato è più cauto, è un danno minore, una modalità di scelta di un capo meno appariscente del presidenzialismo. È possibile che per qualcuno della maggioranza questo metodo di scelta del capo sia meno appariscente. Questo però non esclude assolutamente che sia meno pericoloso sul piano degli equilibri, dei pesi e dei contrappesi, della limitazione dei poteri, della democrazia costituzionale. Tutto dipende da come lo fai, questo presidenzialismo, da come fai questo premierato. Se la forza del premierato trova le sue basi sulle ceneri degli altri poteri, se va ad incidere sulle competenze più incisive, se limita le funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica, assolutamente diventa pericoloso e quindi non costituisce assolutamente un danno minore. Questo premierato, il vostro premierato, rincorre il rafforzamento dell'Esecutivo, vuole evitare fastidi, lungaggini, rallentamenti. Non disturbare chi vuole fare, diceva Giorgia Meloni; ora capiamo a chi si stesse riferendo. Capocrazia con contrappesi che saltano. È pericoloso. Quello che si vuole è una forma di Governo che ricorda un po' quello desiderato da altri in passato. Vi vado a leggere un estratto di un importante dibattito: «Un Governo nella sua più alta, ma anche più concreta significazione d'istituto, atto a risolvere nel modo più rapido, fermo, univoco tutte le molteplici questioni che nell'azione quotidiana si presentano, non impacciato da preventive compromissioni, non impedito da divieti insormontabili, non soffocato da dissidi». L'autore di questo passo è Mussolini, nel dibattito sulla legge Acerbo: ecco perché voteremo a favore di questo emendamento. *(Applausi)*.

va bene. Vorrei indurre alcuni colleghi della maggioranza a riflettere su un fatto. Credo che sia nell'interesse di tutti favorire la crescita economica del Paese e favorire gli investimenti. Vi faccio allora una domanda: quale imprenditore investirà mai in un Paese in cui la stabilità viene riposta sugli umori di una sola persona? Vi chiedo, colleghi: quale imprenditore investirà mai in un Paese in cui, se questa persona si dimette, può far sciogliere le Camere e quindi, se cade il Governo, cade anche il Parlamento? Altro che stabilità. State vendendo un'illusione di stabilità, quando in realtà create un'instabilità più grande. Confidate soltanto sul fatto i parlamentari faranno magari una scelta opportunistica, cioè privilegeranno una scelta conservativa piuttosto che sfiduciare un *Premier*, sapendo che, se lo sfiduciano, poi dovranno tornare a casa. Uno degli auditi ci stava dicendo che una volta i matrimoni erano stabili, perché non c'era la legge sul divorzio. Erano stabili, ma non erano matrimoni felici. Qui si rischia di creare delle accozzaglie di programmi semplicemente funzionali ad avere i numeri per governare e per avere la maggioranza, senza una visione comune sul futuro dell'Italia. Diventa uno scambio di di capricci, come uno scambio di capricci è stato quello che si è visto in questa maggioranza: da un lato un'autonomia differenziata che vuole decentrare il potere, dall'altro un presidenzialismo che lo vuole concentrare su una sola persona. Un altro Gruppo ha voluto mettere le mani su una riforma della giustizia. Oltretutto, parlando di imprenditoria, benissimo: sapete che gli imprenditori vogliono avere anche un contesto di legalità? E voi come combattete la corruzione? Rendendo più difficili le intercettazioni? Questo è il modo in cui volete favorire la crescita economica del Paese? E come pensate di risolvere il problema delle aree di crisi industriale complessa? Guardate che qui non stiamo parlando del Sud Italia. Le aree di crisi industriale complessa si trovano in tante Regioni italiane, comprese quelle del Nord, e in molti casi gli investimenti non vengono fatti in quelle aree perché ci sono delle carenze infrastrutturali. Come glielo dite a quegli imprenditori che nella riforma sull'autonomia differenziata avete bocciato gli emendamenti che prevedevano la perequazione infrastrutturale? Colleghi, se lo Stato ha sempre e solo investito in alcune aree del Paese nelle infrastrutture, creando le condizioni per la crescita per lo sviluppo, vogliamo creare le stesse condizioni anche nelle altre prima di parlare eventualmente di autonomia differenziata? Parliamo di autonomia differenziata, ma sapete che vi è anche la certezza del diritto e se un imprenditore vuole avviare qualche attività in più Regioni, deve avere a che fare con normative diverse da una Regione all'altra? Vi rendete conto che è una follia? Parliamo della certezza del diritto, di ambiente di legalità: voi dimostrate di non avere idea di cosa è necessario per l'Italia. State distraendo le masse, state cercando di fare leva sulle loro paure, perché l'unico obiettivo oggi che avete è andare verso una forma di potere autoritario: fare a meno del Parlamento per avere le mani più libere, cosa che state già facendo, perché lo state dimostrando attraverso questo abuso costante della decretazione d'urgenza.

per cause diverse dalle dimissioni. Succede in realtà che il Presidente del Consiglio avrebbe l'opportunità di decidere di dimettersi, calcolando il fatto che le dimissioni siano a seguito di un periodo inferiore ai due anni e quindi garantirsi

buonafede, nella buona predisposizione e nell'onestà del Presidente del Consiglio. Visto però che non sappiamo chi sarà il Presidente del Consiglio, visto che non sappiamo se il Presidente del Consiglio conduca a una deriva autoritaria o impazzisca, direi che questa è una norma di buonsenso. Del resto, stiamo cercando di legiferare sulla Costituzione, quindi dobbiamo essere prudenti; il principio di precauzione è quello che deve prevalere, quindi dobbiamo prendere in considerazione tutte le possibilità, tutto tutto quello che potrebbe accadere. Non mi sembra prudente non prevedere il fatto che il Presidente del Consiglio potrebbe essere meno onesto di quanto uno confidi che sia. La nostra è una norma prudenziale e, secondo me, è pericoloso che il testo venga licenziato senza paracadute. Purtroppo in quest'Aula siamo in una situazione ridicola, nel senso che l'opposizione continua a rappresentare le proprie osservazioni, ma la maggioranza

voi parlamentari della maggioranza. Avete ricevuto dal vostro capo l'indicazione di un comportamento e vi attenete a quello che il vostro capo vi ha detto di fare, senza usare il vostro cervello, senza usare il vostro spirito critico.

il Senato e la Camera dovessero essere l'espressione popolare delle persone in carne ed ossa, con una rappresentazione proporzionale dei cittadini e delle cittadine.

senza spiegare come sarà la legge elettorale, ma di per sé è una legge di trascinamento: teoricamente si potrebbe prendere il

Qui non potete dire che forse introducete il doppio turno; a parte questo, però, il dibattito è che uno è eletto Presidente quando ha ottenuto la maggioranza più uno dei voti o quando è primo rispetto a un numero

è per questa ragione principalmente che siamo totalmente contrari. Certo, abbiamo presentato emendamenti ostruzionistici per questa ragione: bisogna fare in modo che davvero cerchiate di ascoltare, perché non è che quello che si dice dall'opposizione sia vangelo, ma neanche quello che dice la maggioranza lo è. In Parlamento la discussione è fatta per tener conto ovviamente delle opinioni, anche perché le le regole valgono per tutti: oggi siete in maggioranza, ma domani potreste essere all'opposizione,

dove si gioca; si può vincere e si può perdere, ma le regole devono essere condivise e voi fate una legge che non è condivisa, questo è il dato.

da quando avete deciso di applicare il canguro, abbiamo chiesto di conoscere in anticipo i criteri che la Presidenza decide di seguire. accorpati più di 60 emendamenti e lei, a differenza delle precedenti Presidenze, non ci ha neanche detto fino a che pagina quel voto avrebbe determinato di giungere. Allora, è un problema di rispetto delle prerogative dei senatori. C'era una serie numerica, però il Presidente del Senato lo aveva già chiarito tre volte in Capigruppo, quindi magari può parlare col suo Capogruppo. Passiamo a pagina 350, all'emendamento 5.1668. Scusi, lei sta parlando senza microfono, quindi non viene registrato: se vuole ridirlo, le do la parola. Procediamo o vuole parlare? Presidente,

un Gruppo o un senatore possono decidere di fare una dichiarazione di voto su un emendamento che sa che verrà precluso. Nel momento in cui lei non lo fa in anticipo, noi ci troviamo a 60 pagine di differenza e non possiamo più fare la dichiarazione di voto su un emendamento che verrà precluso. *(Applausi)*. Non è un modo di procedere ed è solo lei che sta procedendo così, perché gli altri Presidenti fino adesso hanno proceduto in maniera corretta, cosa che lei non sta facendo. Va bene, era una serie numerica, ma da ora lo faremo tutte le volte. Così

perché immagina che così il tempo scorre e quindi le prerogative delle opposizioni si riducono. Io non credo che questo sia un modo particolarmente elegante di garantire il confronto su una riforma così significativa: pensare che, facendo valere quelle che sono, a nostro avviso, gravissime scorrettezze procedurali, si riduca la possibilità di intervenire sul merito. Signora Presidente, il nostro Capogruppo non è a conoscenza di come la Presidenza intenda accorpare gli emendamenti e applicare il meccanismo del canguro. Io non so se lei fa riferimento a una qualche comunicazione della Conferenza dei Capigruppo. A noi non risulta che ci sia stata nessuna determinazione della Conferenza dei Capigruppo che ha definito, in via generale e astratta, i criteri di applicazione del meccanismo Per un gesto di riguardo nei confronti dell'Assemblea, chi presiedeva fino ad oggi anticipava quali erano i criteri o almeno anticipava il numero degli emendamenti da accorpare. Il fatto che lei abbia risposto invitandomi a parlare col mio Capogruppo e adesso sorrida di fronte al fatto che noi stiamo impiegando del tempo che va a detrimento della possibilità di intervenire sul merito la dice lunga su come la maggioranza intende aprire un confronto sulla riforma costituzionale. *(Applausi)*. Signora Presidente, mi lasci anche dire che io trovo curioso che, dopo un'intera giornata di dibattito sull'articolo che rappresenta il cuore della riforma, perché è l'articolo che prevede l'elezione diretta la ministra Alberti Casellati non abbia sentito il dovere di prendere la parola e spiegare perché questa riforma risolverebbe i problemi di stabilità e, soprattutto, quale sia la legge elettorale che consentirà alla riforma di essere applicata in maniera conforme a quei principi che pure, ogni tanto, il Governo dice di voler rispettare. Che su un articolo così il Governo e la maggioranza non sentano il dovere di intervenire e spiegare le proprie ragioni, io lo trovo veramente avvilente per la serietà di questo confronto.

indurre a una riflessione su un fatto che secondo me è fondamentale: se volete l'elezione diretta del *Premier*, perché non la staccate dall'elezione del Parlamento? elezioni separate. Se il *Premier* si dimette, perché deve crollare anche il Parlamento? I cittadini esprimeranno di nuovo la loro volontà sul nuovo *Premier*, perché magari in quel momento non sono cambiate le maggioranze, il *Premier* può avere mille ragioni diverse per dimettersi. Voi gli state dando questo potere enorme di dimettersi e di far tornare tutti a casa quando non ce n'è bisogno. Volete l'elezione diretta? Benissimo, ma prevedete un'elezione separata, magari la terrete contestualmente o il mese dopo, ma non potete

ai cittadini e continuate a vendere l'illusione che si tratti solo di scegliere il *Premier*. La presidente Meloni ha fatto un video dove finge di non sapere oppure non conosce questo provvedimento, perché continua a dire che si tratta soltanto di eleggere il *Premier*, non dice che si tratta di una modifica della Costituzione, di un attacco alle cariche istituzionali, come quella del Presidente della Repubblica, di una marginalizzazione del Parlamento che non conterà più nulla. Non dite quali sono i reali contenuti, state facendo vedere soltanto una parte minimale, soltanto la prima riga di un articolo di una riforma che invece soppianta la nostra Costituzione e i suoi valori portanti. A questo punto

dagli studi giuridici, dai manuali di diritto, ed esiste il diritto costituzionale per sentito dire. Se parliamo di diritto costituzionale, dobbiamo anche sapere che cosa è lo Stato di diritto. Se parliamo di Stato di diritto, dobbiamo sapere che è un valore fondamentale non soltanto per l'Italia, ma per l'Europa intera. Se parliamo di Stato di diritto, dobbiamo sapere che lo Stato di diritto è anche la separazione dei poteri, se sappiamo cos'è la separazione dei poteri, sappiamo anche che è la garanzia del sistema democratico. prenda una volta per tutte la parola e ci spieghi come pensa di garantire lo Stato di diritto e la separazione dei poteri con questa riforma.

pone un tema nodale rispetto alla questione dell'equilibrio dei poteri e alla questione legata all'equilibrio elettorale a cui facevo riferimento anche nei precedenti interventi. Abbiamo posto, in sede di dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti, il tema della introduzione di un meccanismo equilibrato per l'elezione diretta del *Premier* abbiamo fatto l'esempio della proposta del costituzionalista Duverger, che introdusse questa discussione nell'ambito della riforma della Quarta Repubblica francese, che poi portò al meccanismo di cui il presidente Macron si è avvalso e che farà scattare l'elezione dell'Assemblée nationale nei prossimi giorni. È evidente che c'è una separazione tra l'elezione del Presidente della Repubblica e l'elezione dell'Assemblea nazionale, che sono due cose distinte e in un caso vi è una attribuzione specifica che, per questo motivo, vede un'elezione distinta. Ora, non è scandaloso immaginare un meccanismo di questo tipo. Serve un impianto di coerenza che non c'è all'interno della norma che il Governo mantiene. Appare Appare quindi di tutta evidenza che serve recuperare questa coerenza di sistema che c'è in Francia, che ci dovrebbe essere anche in Italia e questo ci porta a votare a favore di questo emendamento perché introduce esattamente quell'equilibrio fra il Parlamento e un *Premier* eletto direttamente dai cittadini e consente di fare un'operazione che questa proposta di riforma invece non intende realizzare.

Presidente, fa il suo lavoro: c'è un canguro in ballo e di conseguenza, se gli emendamenti ne racchiudono altri, è chiamata a dirci quali pagine saltiamo e quindi quali parti vengono saltate. Non me la sto prendendo con lei, però mi chiedo,

gli astenuti in Italia sono stati tantissimi, perché alla fine il risultato è che neppure chi è dentro il Parlamento è interessato alle cose che si stanno facendo.

commenti. Avendo gli occhiali e leggendo i labiali, riesco a capire che cosa viene detto. Non volevo sicuramente mancare di rispetto alla Presidenza rivolgendomi direttamente ai colleghi dell'Aula. L'articolo 5 nasce da una rivisitazione totale e complessiva per opera del Governo attraverso un nuovo emendamento rispetto al testo che era stato presentato inizialmente. È questo il motivo per cui noi abbiamo presentato così tanti emendamenti

Il motivo per cui l'articolo 5 è così ricco è perché noi lo riteniamo il cuore del provvedimento. l'articolo che toglie sostanzialmente qualsiasi potere agli eletti dei cittadini. Li toglie

il Parlamento e, in questo modo, toglie la possibilità ai parlamentari di poter svolgere il loro lavoro di eletti. eletti. Presidente, lei ha esperienza anche di Capogruppo e di gestione dei gruppi parlamentari e sa che, per esempio, quando si fanno le riunioni all'interno di una maggioranza che sostiene un Governo

magari vorrebbe agire diversamente e dunque si pone sul tavolo della discussione, legittima e dialettica, il valore che ciascuno di noi si porta dietro. In questo modo tutta quella parte, tutta quella discussione e tutto il lavoro di mediazione che poi dovrebbero riproporsi in Assemblea vengono assolutamente eliminati perché

parlamentare. Presidente, noi continueremo sull'articolo 5, perché esso metta al centro il Parlamento. A voi del Parlamento non interessa, noi lo difenderemo con gli strumenti nelle nostre mani, in questo caso gli emendamenti che seriamente abbiamo presentato.

Signora Presidente, questo articolo è il cuore della riforma della Costituzione. Qui state inserendo il premio di maggioranza in Costituzione, senza aver dato a questo Parlamento neanche la minima idea di come sarà la legge elettorale. Ora, io capisco che voi siate persone perbene e che quindi farete una legge elettorale

far cambiare idea o che possa essere utile a un dibattito. Quindi, Presidente, la invito a chiedere al suo Gruppo (Forza Italia) di resuscitare la proposta di Berlusconi di far votare solo i Capigruppo, in proporzione alla presenza in Aula del Gruppo. Tanto una stupidata già la state facendo: portatela fino in fondo, fate votare solo i Capigruppo e sarete a posto, tutti felici e contenti. Signora Presidente, è troppo importante quello che stiamo discutendo per per non tentare sino all'ultimo di far cambiare questa idea malata di stravolgimento della nostra Costituzione che è nel provvedimento. Nonostante Nonostante tutto il dibattito che c'è stato in Commissione, ampio e profondo, quello che stiamo verificando in Aula è un atteggiamento di chiusura totale, per cui ogni emendamento deve essere sempre respinto. Se abbiamo ancora, Presidente, un po' di senso di dignità del ruolo, è evidente che il sistema che si propone non ha riferimenti e paragoni in nessun altro Paese. L'unico esperimento che c'era stato in Israele, un po' di anni fa, è stato immediatamente superato, abrogato e tolto per il cattivo funzionamento degli organi istituzionali. Perché ostinarsi a non volersi confrontare su un tema così importante che interessa la vita democratica del Paese? L'abbiamo sottolineato in tanti modi: non abbiamo preclusione a discutere un nuovo modello, quello che non è possibile è superare e mortificare una Repubblica parlamentare. Si tolgono le competenze e le prerogative del Presidente della Repubblica e si umilia un Parlamento e, dentro il Parlamento, gli uomini e le donne elette dai cittadini e dalle cittadine. Perché tutto questo? Perché non immaginare che un atto riformatore così importante che cambia il modello, cambia gli assetti istituzionali, cambia i poteri, non si possa fare a botte di maggioranza, ma prefiguri un dialogo diverso, molto profondo, rispettoso, tra maggioranza e opposizione? Il Parlamento a trascinamento che deve il suo destino solo ed esclusivamente alla figura del *Premier* o della *Premier* è un Parlamento che è assoggettato, non è più libero. Non è il Parlamento che prefigura la nostra Costituzione per la quale i Padri e le Madri costituenti hanno trovato un livello di intesa altissimo. Ecco, Presidente, perché continuiamo a batterci per farvi cambiare idea, perché l'idea che avete mina l'idea che avete mina profondamente la nostra Costituzione e il rapporto tra cittadino e istituzione, un cittadino che viene umiliato esattamente come il suo Parlamento. Signora Presidente, prima di qualche osservazione rispetto al tema generale e all'articolo 5, forse l'unica cosa che condividiamo tra quelle che abbiamo sentito oggi è che l'articolo e l'elemento fondante di questa riforma. Parto però dalle osservazioni della senatrice Furlan, che diceva, Presidente, che questa

bella anche per quello che significa e rappresenta: «Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto». Bene, stiamo ascoltando una serie di interventi che ci vogliono convincere (noi più li sentiamo e più ci convinciamo del contrario, non è che non vi ascoltiamo) vi ascoltiamo) che in queste due righe si nasconde un indebolimento della democrazia; addirittura, in alcuni casi, forse il tradimento della Costituzione. sì, è vero che le riforme si deve cercare di farle insieme, ma quando si confrontano due visioni così diametralmente opposte, arriva pure il momento in cui si deve andare avanti. non riusciamo a comprendere come possa essere più democratico un Parlamento nel quale, solo per fare qualche esempio con riferimento anni, viene nominato un senatore a vita che il giorno dopo diventa Presidente del Consiglio senza essere stato eletto dai cittadini o nel quale, qualche anno dopo uno, un avvocato sconosciuto che non si candida neanche alle elezioni diventa Presidente del Consiglio. Noi pensiamo che sia più democratico lasciare ai cittadini questa scelta *(Applausi)* e crediamo che questo non interferisca in nessun modo con le prerogative del Parlamento con le prerogative del Parlamento e con il ruolo del Presidente della Repubblica, che in questa proposta viene confermato e che resta arbitro e garante delle Istituzioni, come è giusto che sia. abbiamo ascoltato, ma ci avete sempre più convinti di quanto sia giusta la strada che vogliamo intraprendere. *(Applausi)*. Ci siamo convinti sempre di più che questa riforma rafforzerà la democrazia e non la indebolirà. A questo punto, è nostro compito andare avanti e saranno i cittadini, come la Costituzione stessa prevede, a decidere se ritengono giusto questo intervento, a fare in modo che la sovranità popolare, i cui limiti sono modificabili dalla stessa Costituzione (che prevedeva di poter essere modificata nel suo assetto), sia determinabile fino in in fondo e se possa essere quindi lasciata ai cittadini questa scelta. Noi siamo convinti che sia giusto così e alla fine saranno i cittadini stessi a decidere. Signora Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento, esattamente per le motivazioni che ha spiegato il senatore De Priamo, che ha fatto una *consecutio* illogica rispetto alla sua premessa.

è questo quello che contestiamo della vostra riforma. Il Presidente francese scioglie le Camere, che vengono elette in un momento separato da quando viene eletto lui; le due cose sono scisse: è esattamente quello che vi stiamo dicendo da mesi. Non potete fare le due votazioni insieme, perché non c'è bilanciamento tra i due poteri. Allora decidetevi: se vi piace il modello francese, scegliamo il modello francese, ma non è quello che ci state proponendo voi. Voi mettete mettete insieme capre e cavoli; mettete insieme potere esecutivo e potere legislativo. *(Applausi)*. Voi volete, neanche con due schede ma con una sola scheda, mettere insieme di due poteri che la nostra Costituzione tiene ben separati. Fate pace con la logica: o l'uno o l'altro. *(Applausi)*. Tutto insieme è un minestrone, non va

paragoni logici. Se volete difendere questo pastrocchio, almeno trovate un paragone logico che sia uguale. Ma non lo trovate perché sul globo terracqueo

questa proposta e ovviamente noi cercheremo di contrastarla democraticamente in Parlamento. Già da adesso organizzeremo i comitati con cui chiederemo di bocciare questa riforma costituzionale. Intanto

che toglie i poteri al Capo dello Stato, mettendo in discussione la Costituzione, nata - e vorrei sottolinearlo senza provocare - dalla lotta della Liberazione e della Resistenza, quindi

questo è il dato fondamentale. Il problema allora è che il Parlamento dev'essere libero ed eletto dai cittadini e dalle cittadine in modo democratico: voi questa cosa non la state facendo. Inoltre, non spiegate quanto è il premio di maggioranza.

come dev'essere questa legge elettorale e quindi a quanto ammonta il premio di maggioranza; nello stesso tempo legate l'elezione del *Premier* all'elezione dei deputati e dei senatori. In questo caso,

perché è stato eletto, per trascinamento - intrinsecamente è meno libero, perché questo sta nella natura della persona umana, non so come spiegarlo. Questo è il dato fondamentale: cerchiamo almeno di evitare queste cose, in modo tale di sostenere le proprie opinioni senza avere il timore, come si dice, di essere messo alla berlina, perché in sostanza c'è qualcuno che decide al suo posto.

convocata per le ore 20,30, quindi chiederei che i lavori si interrompessero in tempo, perché il mio Gruppo possa partecipare, quindi con un'interruzione alle ore 20,15 o alle 20,20, in modo da consentire insomma al mio Gruppo di partecipare a questa riunione. Senatrice Maiorino, come sapete tutti, oggi la seduta non prevedeva un orario di chiusura, ma, proprio su richiesta del suo Capogruppo, il presidente La Russa ha concordato un orario di chiusura per le ore 20,45. Quella è stata un'interlocuzione del tutto informale, avvenuta tra il presidente La Russa e il presidente Patuanelli, però faccio presente che la riunione del mio Gruppo inizia alle ore 20,30, quindi, francamente, abbiamo trovato la concessione delle ore 20,45

Presidente, non vorrei che diventasse prassi il fatto che ci sono degli accordi che non vengono sottoscritti. È già la seconda volta che accade oggi. Io non sono voluto intervenire in precedenza, perché il livello e lo spessore della figura che veniva ricordata, quella dell'onorevole Enrico Berlinguer, non dovevano essere sporcati in alcun modo da una polemica di carattere procedurale. Posso solo dire che avrei voluto portare, a nome del mio Gruppo, un momento di omaggio alla memoria e al ricordo dell'onorevole Berlinguer. Nella circostanza, però, noi abbiamo appreso in Aula abbiamo appreso in Aula che era intercorso un accordo fra uno o più Gruppi e il Presidente e il Presidente, *motu proprio*, ha ritenuto di circoscrivere il dibattito, come è avvenuto. Noi ne abbiamo preso atto,

presiedo un Gruppo, ma nessuno mi ha chiesto nulla e tantomeno abbiamo concordato nulla. Basta chiedere e si ha una risposta, ma che non diventi una prassi che si parla con uno e questo significa che tutti sono d'accordo. Vale per gli interventi di prima, vale per l'orario di chiusura, varrà domani per altre questioni. a prescindere dal fatto che vi siano state delle interlocuzioni formali o informali, a noi sembra che la richiesta della senatrice Maiorino sia da sostenere. Noi la sosteniamo, anche perché significherebbe chiudere solo quindici minuti prima dell'orario di chiusura previsto. Mi sembra una richiesta di buonsenso che, peraltro, è sempre avvenuta su richiesta dei Gruppi.

io qui vorrei commentare il fatto che si dicono cose a sproposito, a testimonianza di quello che diceva la senatrice Malpezzi, non si sa cosa si vota e, purtroppo, non si sa nemmeno cosa si dice a proposito dell'Inghilterra. È vero che il primo ministro Sunak ha chiamato le elezioni, ma quando si è dimesso Boris Johnson, il Parlamento non si è sciolto. Le due cose sono completamente distinte. Vorrei dire ancora una cosa in proposito. In Inghilterra ci sono 785 senatori a vita che siedono nella House of Lords

Adesso, per sciogliere il Parlamento, bisogna chiedere il permesso al re. Si chiama *royal prerogative*. Quindi, vi chiedo, prima di dire stupidaggini, di pensarci.

Signor Presidente, ora ho capito perché non intervenite: perché tutte le volte che interviene qualcuno della maggioranza dice un sacco di fregnacce.

È chiaro ed evidente che non è che siete solo così, voi siete pericolosi, siete estremamente pericolosi perché non sapete cosa state facendo. Questa riforma cosa fa? Sposta tutto il potere legislativo sotto l'Esecutivo, depotenzia il Presidente della Repubblica, togliendogli il ruolo di equilibratore del sistema

MARTON *(M5S)*. Il disegno ai cittadini è chiaro: potere legislativo non più al Parlamento, che viene esautorato totalmente; parlamentari eletti a strascico del Presidente del Consiglio, che avrà potere di vita e di morte sul Parlamento; tutta la parte legislativa sotto una sola persona; Presidente della Repubblica che non ha più potere di fare alcunché perché è obbligato a sciogliere le Camere sulla base dei *desiderata* del Presidente del Consiglio di turno. Voi non siete a posto, io ve lo dico.

forti ed alti principi costituzionali, bisognerebbe evitare il turpiloquio e gli insulti. Questo farebbe salire il livello. Siccome c'è stato un intervento del senatore De Priamo che è stato definito dal precedente intervento - al di là delle parole del tutto inappropriate -

il Presidente del Consiglio sfiduciato può chiedere lo scioglimento del Parlamento, ma può anche non chiederlo, per cui è esattamente la stessa cosa. Quanto al fatto di comunicarlo al re, vorrei al re, vorrei sapere se sa citarci un caso nella lunga storia dell'attuale assetto costituzionale - so bene che non c'è una Costituzione, ma loro lo chiamano *constitutional*, lo dico per evitare che poi qualcuno dica che non so che non c'è una Costituzione scritta cui il re o la regina si siano rifiutati di sciogliere il Parlamento quando il Primo Ministro l'ha chiesto. La risposta è facile, perché non è successo mai. I paragoni, quindi, sono del tutto appropriati. È vero che l'Italia è diversa da ogni altro ordinamento di altri Stati e dunque non c'è nulla di strano che anche questa riforma sia diversa da quella degli altri Stati, perché ad esempio con il cancellierato alla tedesca

il Primo Ministro inglese doveva chiedere il permesso alle Camere per sciogliere il Parlamento. Dal 2022 questo diritto è ritornato al re, punto e basta. Questa è la legge inglese, studiatevela.

Signora Presidente, ho appena telefonato al Re d'Inghilterra, che mi ha detto che Sunak ha deciso autonomamente di fare le elezioni e che non ha chiesto il permesso al re. Me lo ha detto l'amico Carlo, grazie.

Presidente, interveniamo su questi grappoli di emendamenti che vengono mangiati dai canguri soltanto per dire che, al di là del contenuto del singolo emendamento, di richiamare il Governo a un'attenzione alle indicazioni che dovranno essere date a queste Camere su come funzioneranno il premio di maggioranza e la legge elettorale. Gli emendamenti che stiamo votando sono stati cioè presentati per richiamare il Governo e la maggioranza a un'attenzione circa la rilevanza costituzionale che assume la legge elettorale e quindi la necessità che questo Parlamento voti consapevolmente sapendo quale sarà il meccanismo, quale sarà il premio di maggioranza e come funzionerà, perché costituzionalizzando questo meccanismo, se non sappiamo quale sarà il suo contenuto, ci chiedete di votare alla cieca su un testo che fondamentalmente rimanda al nulla.

lei immagina di definire la legge elettorale, prevista dall'articolo Vada pure avanti, senatore Giorgis. come il Governo e la sua maggioranza immaginano di applicare questo articolo 5 nella parte in cui prevede espressamente che la legge elettorale garantisca garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del

alle liste, qualora le liste collegate dovessero raggiungere una maggioranza intorno al 25 o al 30 per cento. Perché le rivolgo questa domanda? Innanzitutto perché così noi potremmo sapere di che cosa stiamo discutendo - vale per l'opposizione, ma a maggior ragione per la maggioranza - e poi perché, se non ricordo male, sia lei che il relatore, in Commissione e in Aula, avete fatto cenno all'ipotesi che la legge elettorale che intendete proporre ipotizzi la soglia di consenso necessario per far scattare il premio al 40

quei principi che la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito in base ai quali non è costituzionalmente legittimo attribuire dei premi che determinano una disproporzionalità tale da trasformare una minoranza in una consistente maggioranza. Poco tempo fa il senatore Priamo si è alzato e ha replicato alle nostre preoccupazioni e io per questo lo ringrazio.

da mesi in Commissione e non volevo assolutamente mancare di riguardo non citando il nome correttamente e neanche sto parlando con ironia. Sto parlando con rispetto facendo notare all'Assemblea come quando il senatore De Priamo si è alzato e ha finalmente dato voce a una qualche replica, si è aperto in quest'Aula un qualche confronto, un qualche dibattito. Quante ore ci sono volute però perché in quest'Aula si aprisse un momento di confronto? Vorrei allora che domani la Ministra consentisse a quest'Aula di discutere con consapevolezza del significato del testo svelandoci

sollecito questa richiesta che faceva anche il senatore Giorgis, perché è scritto qui in sostanza che si vuole un premio di maggioranza. Io, a differenza di altri colleghi, penso che la maggioranza abbia molto chiaro cosa vuole. Questo è il punto. Lo abbia talmente chiaro che è una scelta politica, quindi io non mi sento di dire che qualcuno non ha capito, non capisce o cose di questo genere. Penso che sia molto chiaro

sotto la tutela di chi lo presiede. Questo è il dato ed è francamente una scelta politica, che potete anche sostenere, però lo dovete fare in modo molto chiaro.

di avere chiaro che cosa volete.

grazie.